il 2 marzo, in occasione delle iniziative «*Senato & Cultura»*, quest'Aula si è tinta di rosa per rendere omaggio alle tante eccellenze femminili, in ogni possibile declinazione artistica. Questa è stata anche l'occasione, per noi, per riflettere, in vista dell'8 marzo, sulla storia dell'emancipazione delle donne: una storia fatta di sacrifici, di lotte ma anche di traguardi, anche di affermazioni e di conquiste. Tuttavia, al di là delle conquiste raggiunte, che sono state tantissime, ci sono, a mio parere, ancora tante cose da fare: penso agli inaccettabili, preoccupanti, casi di violenza; penso, ancora, alle limitazioni di libertà, che ci sono e sono ancora presenti in molti Stati; penso, ancora, alle discriminazioni esistenti in grande parte del nostro pianeta. Ed allora, nella storia delle donne, credo ci siano ancora tante e tante pagine da scrivere e penso anche che voi senatrici, con il vostro impegno, con la vostra passione, con la vostra competenza e con la vostra professionalità, saprete dare a quest'Aula un grande contributo. Consentitemi, allora, di poter offrire un omaggio floreale a voi tutte per celebrare tutti assieme, senatrici e senatori, l'8 marzo. *(Gli

La Conferenza dei Capigruppo ha adottato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 marzo. Nella seduta di oggi si svolgerà la discussione generale sul decreto-legge sulla Banca Carige, il cui esame proseguirà nella giornata di domani. Il calendario della settimana corrente prevede, inoltre, la discussione delle mozioni sull'istituzione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, sulla coltivazione e commercializzazione della canapa e sulle misure per fronteggiare le malattie oncologiche, e - alle ore 9,30 di giovedì 7 marzo - la discussione delle mozioni sul TAV Torino-Lione. Restano confermati gli altri argomenti della settimana incluso il *question time*, per il quale è prevista la presenza dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della pubblica amministrazione e degli affari regionali. La settimana da lunedì 11 a venerdì 15 marzo sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Martedì 19, alle ore 15,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 Marzo 2019. Mercoledì 20 sarà discussa la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti del ministro Salvini. Per consentire di porre ai voti la proposta della Giunta alle ore 13 e organizzare il relativo dibattito

il dibattito potrà pertanto avere inizio anche nella seduta di martedì 19 marzo, dopo la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Il risultato della votazione non sarà proclamato immediatamente,

in un apposito verbale nel prosieguo della seduta, fino alle ore 19. Il calendario di tale settimana prevede, inoltre, il seguito degli argomenti non conclusi, la discussione della mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Toninelli, giovedì 21 marzo, i disegni di legge sul salario minimo orario (ove conclusi dalla Commissione), il sindacato ispettivo e - alle ore 15 di giovedì 21 - il *question time*. Nella settimana dal 26 al 28 marzo l'Assemblea si riunirà per la possibile terza lettura del decreto-legge su reddito di cittadinanza e pensioni e del disegno di legge sulla legittima difesa, quest'ultimo ove concluso dalla Commissione. Saranno inoltre discusse le mozioni sull'autismo e sulle riserve auree della Banca d'Italia. Comunico che la Presidenza ha conferito ai senatori Questori l'incarico di svolgere opportuni accertamenti istruttori relativi a comportamenti tenuti da alcuni senatori, secondo le segnalazioni che sono state sottoposte alla Presidenza, nel corso dei lavori dell'Assemblea e anche

il Partito Democratico ha votato contro il calendario in esame. Avremmo voluto infatti calendarizzare la mozione di sfiducia individuale al ministro Toninelli quanto prima possibile e la nostra proposta era di farlo martedì della prossima settimana. Credo che il ministro Toninelli abbia perseguito con grande determinazione, in maniera davvero molto determinata, la ricerca di questa mozione di sfiducia, visto che ne ha combinate di ogni a danno del nostro Paese e della nostra comunità nazionale.

che porta la calendarizzazione della mozione di sfiducia al ministro Toninelli il giorno dopo - guarda caso, proprio il giorno dopo! - l'esame della richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro Salvini.

5 Stelle cominci a diventare molto pesante per la nostra democrazia e quindi siamo molto preoccupati. Aggiungo che abbiamo chiesto spiegazioni rispetto agli atteggiamenti della maggioranza sulla Convenzione di Faro, perché ci viene dato il contentino di calendarizzarla ogni tanto, ma ogni volta ci si rifiuta di discuterla. La proposta che chiediamo di mettere in votazione, è di inserire per martedì della prossima settimana la calendarizzazione della mozione di sfiducia individuale al ministro Toninelli,

che perderemmo nel caso si mantenesse la posizione di contrarietà alla linea ad alta velocità che colleghi l'Italia alla Francia e non già semplicemente il Piemonte a Lione, come ha sottolineato il Ministro, dimostrando di non avere una grande idea del complesso delle infrastrutture del nostro Paese: è il collegamento dell'Italia con la Francia e con i grandi traffici di merci e di persone a livello internazionale. In altre parole, si tratta nella parte più produttiva, più avanzata, che possa avere maggiori prospettive di sviluppo nel nostro Continente, oppure restare nella parte emarginata. I dati sull'evoluzione del prodotto interno lordo dimostrano che già oggi, grazie a questo Governo, siamo nella parte emarginata. Dobbiamo assolutamente impedire al al Governo di tagliare le gambe al progresso nei prossimi dieci, vent'anni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Dobbiamo avere un centesimo della lungimiranza che ebbe Camillo Cavour negli anni Cinquanta dell'Ottocento, che ebbe quel Parlamento. Per questo abbiamo presentato la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Toninelli; non tanto nei confronti della sua persona, che pure ci ha abituati a una serie di atteggiamenti che ci possono lasciare perplessi, ma per questo aspetto ma per questo aspetto specifico, ossia il suo no, ribadito in tutti i modi e con tutti i pretesti, alla linea ad alta velocità. Abbiamo aspettato mesi per uno studio costi-benefici, i cui

L'unico che non era allineato si è rifiutato di firmare la relazione, perché assolutamente non condivisibile. Poi abbiamo avuto una relazione per cui abbiamo scoperto che questi costi sono comunque trattabili: il costo è 3 miliardi e mezzo, però trattabili, per cui potrebbero essere un po' di meno. Poi si parla del mini TAV, dimenticando che questo è un progetto a livello internazionale, sancito da un trattato internazionale. È una cosa gravissima: fa perdere credibilità all'Italia, ben al di là di là dello specifico fatto della linea ad alta velocità, che pure è importantissimo. Ci interessa di meno il fatto che la discussione della mozione sia prima o dopo il 20 marzo, quando è stabilita la votazione sulla questione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, perché sul perché sul TAV siamo sempre stati a favore, sempre, costantemente, senza rallentare, senza avere una parola a Roma, un'altra a Torino e un'altra in Val di Susa come altri hanno tenuto nella seconda parte della scorsa legislatura ci fosse stato più attivismo sul TAV, oggi saremmo molto più avanti e sarebbe molto più difficile per questo Governo irresponsabile bloccare

in qualunque momento prima del 20 marzo e non perché il 20 marzo si vota sul ministro Salvini, ma perché quella è la scadenza entro la quale l'Italia si deve muovere se non vuole perdere subito, irrevocabilmente, 300 milioni di euro. Poi, qui si porteranno risparmi risibili su altri argomenti, ma intanto si perdono 300 milioni.

a portare a buon fine la ratifica da parte del Parlamento della Convenzione di Faro. Come lei sa, Presidente, ne abbiamo discusso anche oggi: era arrivata in Aula ed è ritornata in Commissione. in Commissione. Francamente, non riesco davvero a comprendere i motivi per cui, da parte della maggioranza - o almeno di una parte della maggioranza - si continui a osteggiare la ratifica di una convenzione molto importante, che tra l'altro è stata sottoscritta

previsto dal nostro Regolamento, di fare una settimana Aula e una settimana Commissione ed è per questo motivo che la prima settimana utile è quella che va

la mozione di sfiducia l'avete presentata voi; avete chiesto voi di discuterla, per quanto ci riguarda avremmo potuto discuterla anche fra sei mesi, a testimonianza che non c'è nessun *do ut des* sul tema. Capiamo che siamo in un momento dove si devono cercare a tutti i costi alchimie di natura politica. Al presidente Marcucci, noto alchimista della politica italiana, auguriamo buona continuazione e buon lavoro: alla prossima, naturalmente, poiché siamo davvero molto curiosi di vedere cosa si si inventerà per la prossima seduta.

sull'errata scelta della data non solo per i motivi prima detti, ma - soprattutto - per l'urgenza che il tema della sfiducia al ministro Toninelli riveste.

La prossima settimana ci sarà una grande manifestazione del settore, colpito da una crisi che ha già determinato la riduzione di 600.000 posti di lavoro. Sarebbe necessaria una seria politica di programmazione e rilancio delle opere pubbliche e, per fare questo, occorre un Ministro competente, cosa che - di tutta evidenza non è il ministro Toninelli. C'è poi una seconda ragione molto più cogente e importante: mi riferisco all'attitudine alla menzogna di molti Ministri e, in particolare, in questo caso, del ministro Toninelli. Nella gestione del *dossier* sul TAV ha mentito più volte. Ha mentito al Paese; ha mentito al Parlamento; ha mentito al Governo di un altro Paese; ha mentito all'Unione europea. Menzogne. Ha spacciato l'analisi costi-benefici per attività innovativa; è una menzogna. Ha detto di aver fermato i bandi; un'altra menzogna (in questo, aggiungo, per fortuna). Ha dichiarato che non esiste alcun *tunnel* scavato in quel posto, evidentemente continuando a fare confusione con quello del Brennero. Quello non esiste, mentre gli altri esistono! Ci sono già diversi chilometri del *tunnel* di base scavati, oltre alle gallerie di servizio. Ha incaricato una Commissione - è stato già detto - tutt'altro che *super partes*. Degli errori dell'analisi costi-benefici parleremo quando discuteremo la mozione. Concludo, signor Presidente, con una questione secondo me delicatissima, ancora più importante e seria. Nell'economia l'affidabilità è un bene primario.

se ogni Governo che arriva cambia le leggi retroattivamente e i contratti e non sta ai patti. Signor Presidente, questo Ministro danneggia gravemente l'economia del Paese e, quindi, i suoi cittadini.

per motivi di salute non potrà svolgere questo compito. Io cercherò di sostituirla in modo adeguato rivolgendole i miei migliori auguri di un pronto ristabilimento. La relazione non presenta particolari asperità, dato che il tema è molto noto sia nelle criticità che sono emerse nella gestione di questo istituto, sia per quel che riguarda l'approccio che è stato adottato, che riprende quello che la precedente maggioranza aveva adottato in alcuni casi analoghi. Ricordo brevemente che le criticità nelle quali è incorso l'istituto hanno

di normative europee che hanno aumentato i requisiti di patrimonializzazione delle banche, portando quindi a successive richieste di ricapitalizzazione. Inoltre, vi sono delle criticità specifiche, delle quali si è ampiamente discusso, che sono riferite alla *governance* dell'istituto in questione, e che, nelle relazioni che sono state effettuate durante le audizioni (il materiale informativo

che sicuramente non hanno aiutato. Il fattore scatenante è stato, come ricorderemo, il fatto che nell'assemblea straordinaria convocata il 22 dicembre 2018 non è stata approvata una proposta di aumento del capitale sociale, che era stata richiesta sulla base di una debolezza patrimoniale rilevata dalla BCE, che aveva chiesto di intervenire. quattro membri del consiglio di amministrazione si sono dimessi e questo ha determinato la decadenza dell'organo. Lo stesso 2 gennaio è stata disposta dalla BCE l'amministrazione straordinaria di Banca Carige, peraltro in continuità sostanziale con l' amministrazione precedente.

e favorire una risoluzione della crisi basata su soluzioni di mercato, come ha esplicitamente affermato il ministro dell'economia e delle finanze Tria nel corso della sua audizione. è diviso in due capi. Il capo I (articoli da 1 a 11) disciplina la concessione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi da Banca Carige (articoli da 1 a 8) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia nel caso si presentino gravi crisi di liquidità, quindi stiamo parlando della cosiddetta Emergency liquidity assistance (ELA). La garanzia naturalmente è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il che significa che è una garanzia garanzia che sostanzialmente si eroga con un costo che deve essere allineato ai costi di mercato. Gli strumenti di debito che possono accedere alla garanzia devono essere stati emessi successivamente entrata in vigore del decreto-legge, essere denominati in euro, avere durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni, prevedere il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza con interessi calcolati sulla base di un tasso costante e predeterminato (cioè essere sostanzialmente a tasso fisso) e poi essere prodotti semplici di tipo *senior*, cioè non avere clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi. La garanzia è onerosa, come già detto, in omaggio alla normativa europea sugli aiuti di Stato, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore degli strumenti finanziari con durata superiore ai tre anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca. Il corrispettivo per la garanzia è differenziato rispetto alla durata dell'operazione con una serie di calcoli, che sono oggetto anche del decreto-legge, e determinato a partire da una valutazione di base che poi è integrata con un componente che misura il rischio di credito riferito a indici di mercato, in linea con le comunicazioni della Commissione. La garanzia deve essere richiesta con una domanda indirizzata al Dipartimento del tesoro e alla Banca d'Italia; quest'ultima ne verifica la congruità e la comunica al Tesoro dopodiché la richiesta di concessione della garanzia viene notificata alla Commissione europea. Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce che la garanzia può essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione. Voglio ricordare, a questo proposito, che nell'audizione della Consob il dottor Apponi, nella sua corposa memoria, ci ricorda che, con comunicato stampa del 18 gennaio 2019, Carige informa di aver richiesto al MEF il rilascio della garanzia pubblica per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di due miliardi di euro, con durata rispettivamente di dodici e La procedura è andata avanti ed è arrivata anche la relativa autorizzazione. Entro due mesi dalla concessione della garanzia, ove le passività non siano già state rimborsate, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia, la Banca Carige SpA è soggetta a vincoli particolarmente stringenti con riferimento alle operazioni che riguardano il proprio capitale: non può distribuire dividendi, non può effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, non può riacquistare tali strumenti né acquisire nuove partecipazioni. Qualora la banca non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita, invia, di norma almeno entro trenta giorni prima della scadenza, una richiesta motivata di attivazione della garanzia alla Banca d'Italia e al Tesoro, il quale provvede al pagamento. La banca rimborsa le somme pagate dallo Stato all'Erario maggiorate con l'applicazione di interessi al tasso legale. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo. poi la garanzia riferita all'ELA, ovvero agli strumenti posti a garanzia della liquidità di emergenza. La garanzia statale, in questo caso, integra il valore di realizzo del cosiddetto collaterale (cioè delle attività finanziarie utilizzate come garanzia per questa erogazione di liquidità) che sia già stato stanziato dal Banca Carige nell'ambito dell'ELA. In caso di inadempimento, la garanzia viene escussa in esito a quella relativa al collaterale stesso per l'importo residuo dovuto. Si applicano, in quanto compatibili, le solite norme relative alla garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione. Il Capo II del provvedimento (che non è ancora stato minimamente attivato) disciplina gli interventi di rafforzamento patrimoniale che consistono nella possibilità di una ricapitalizzazione precauzionale pubblica; a tale scopo viene autorizzato il MEF a sottoscrivere o acquistare azioni di Banca Carige, previa specifica richiesta dell'istituto. Rispetto a tale ipotesi, nel comunicato stampa diffuso l'8 gennaio 2019, i commissari di Banca Carige hanno precisato che le misure di ricapitalizzazione precauzionale sono da considerarsi come misura ulteriore a tutela dei clienti, da attivarsi come ipotesi del tutto residuale. Le richieste di ricapitalizzazione dovranno essere precedute dalla sottoposizione all'Autorità di vigilanza competente di un programma di rafforzamento patrimoniale e questi piani di ristrutturazione dovranno adeguarsi ai principi che la Commissione europea stabilisce, in particolare gli interventi di cosiddetto *burden sharing*, cioè di condivisione di condivisione del peso dell'intervento, ovvero di riparto degli oneri tra obbligazionisti e azionisti. Mi avvio rapidamente a concludere, anche perché vedo che il tema è ampiamente noto e anche abbastanza poco interessante per la maggior parte dei colleghi.

subordinati in circolazione, che in questo caso sono stati sottoscritti dallo Schema di intervento volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi e, per una parte residuale, da Banco Desio nello scorso novembre. Quindi non ci sono investitori *retail* in possesso di strumenti che possono essere convertiti in azioni. Concludo ricordando che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito l'articolo 21-*bis*, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge.

Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, le norme europee, come ha detto il relatore Bagnai, dettano le procedure a tre *step*: garanzia dello Stato su obbligazioni, procedura già attivata per 2 miliardi (due emissioni per un totale di 2 miliardi a dodici e diciotto mesi); il secondo *step* è la garanzia sui prestiti della Banca d'Italia; il terzo *step* è la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dello Stato (procedura già seguita in altri casi).

Come sarà fatta nel piano industriale la valutazione dei titoli dell'attivo? Al valore attuale o al valore di rimborso? La differenza è infatti notevole. Le razionalizzazioni già annunciate attraverso la chiusura di filiali - pare cento magari nei periodi in cui Berta filava, quando non si teneva conto dei costi e dell'antieconomicità di alcune di esse - oppure i mille licenziamenti: questa è la razionalizzazione? Lo dico da forzista liberale: sono contrario. Il recupero della redditività in dodici o diciotto mesi, per restituire il prestito obbligazionario con interessi e una commissione, potrà essere sopportato dalla forbice tra tassi attivi e passivi, oggi molto bassa? sopportate le commissioni bancarie praticate oggi con una certa facilità? Si racconta al mio Paese che un mattino in cui nella banca non c'erano clienti, un impiegato fece all'altro:

che costano, perché vanno spesate nel conto economico (anche se tenendo conto della nascita degli NPL, a due o a sette anni).

in maniera equa, ma tendenzialmente al ribasso, dato che oggi il mercato è al ribasso anche per i *manager*. Potremo mai vedere l'elenco dei debitori più importanti? Lo abbiamo chiesto noi di Forza Italia con un emendamento che probabilmente sarà cassato. Sui controlli di Banca d'Italia e Consob abbiamo assistito alle audizioni congiunte con la Camera, però un ente racconta la storia e getta la responsabilità a carico dell'altro. Credo che sulle banche il controllo debba essere effettuato prevalentemente nel merito da parte di Banca d'Italia. Il Governo vuole nazionalizzare un futuro, attraverso la sottoscrizione del capitale - nella maniera necessaria, ma anche superiore al 50 per cento - oppure è favorevole alle aggregazioni?

avrebbe potuto dire «pago subito il credito d'imposta e non devo neanche fare il prestito; erogo e do la liquidità necessaria all'istituto affinché possa andare avanti»? Si sarebbe

ovviare. Parlo dei nostri emendamenti ed eventualmente anche di altri, di qualsiasi partito: si sarebbe potuto tenere conto di qualche apporto costruttivo, per inserire altri elementi che riguardassero le banche all'interno di un decreto-legge che parla delle banche. Io ho presentato

alle BCC tutti i giorni, *à gogo*, che dettano le future regole, e che le BCC abbiano cominciato a capire che hanno decretato la loro morte. Inoltre, c'è un'azione legale di Cassa Centrale Banca nei riguardi di ICCREA, sulla percentuale superiore al 15 per cento posseduta dai soci di Cassa Centrale in ICCREA, essendo soci pure della stessa ICCREA. La norma prevede il massimo del 15 per cento; quello che è in più deve essere ceduto e non ha diritto di voto. Quindi abbiamo cominciato a creare dei problemi, perché non siamo stati coraggiosi nel mantenere l'autonomia e la mutualità delle BCC. Forza Italia pertanto fatto queste osservazioni, che credo siano, se non condivisibili, almeno accettabili dal punto di vista strettamente razionale e tecnico. al secondo passaggio, ma ci atterremo a questa regola, costruttiva come sempre, su una materia delicata come quella delle banche.

il decreto-legge che quest'Aula si appresta a convertire in legge è intervenuto in un contesto emergenziale senza precedenti e risponde a una prospettiva europea discutibile. In particolare, l'atto di commissariamento del 2 gennaio 2019 ordinato dalla Banca centrale europea, considerato nel dibattito pubblico alla stregua di un atto dovuto, rappresenta il primo di una serie di criticità a livello europeo su cui il Parlamento italiano è chiamato a discutere e a riflettere. Il caso di Banca Carige, infatti, è il primo atto di amministrazione straordinaria disposto da una banca privata qual è la Banca centrale europea, la quale, seppur partecipata dalle banche centrali dei Paesi membri, è indirettamente a larga partecipazione privata. Segue pertanto domandarsi: come è possibile che nessuna istituzione preposta non ravvisi nell'atto di commissariamento disposto dalla BCE un possibile conflitto di interesse, che peraltro può indirettamente favorire qualcuno e svantaggiare altri? Ciò soprattutto laddove la BCE giustifica il provvedimento per la mancata delibera assembleare di portare a patrimonio un debito di 320 milioni, trascurando però le inevitabili ripercussioni che tale decisione avrebbe sul valore di ciascuna azione. Quanto accaduto per Banca Carige si inquadra in una prospettiva più ampia e perversa, praticata ormai da anni, ovvero quella di sostenere, contrariamente alla visione economica americana, che anche le piccole banche In questo ambito, infatti, è venuta a maturare in Italia anche la recente e assurda riforma del credito cooperativo, che tenderà a far scomparire le casse rurali, che da secoli rappresentano per il nostro Paese una forte leva di sviluppo delle economie territoriali. Anche su questa contrapposizione di natura economica la politica dovrà interrogarsi e riflettere, consapevole che, in assenza di un cambiamento radicale, lo scenario bancario è destinato a caratterizzarsi in un futuro non molto lontano per la presenza di poche grandi banche, con inevitabili ripercussioni sull'economia reale per le difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle famiglie. Così facendo, il mercato bancario è destinato all'oligopolio. La problematica di Banca Carige, relativa alla mancata ricapitalizzazione, permette, inoltre, di evidenziare un'altra anomalia del modello bancario europeo, ovvero quella delle regole contabili di valutazione. A tal riguardo, sono state introdotte delle discutibili e rigide regole contabili che prevedono vincoli di natura patrimoniale sugli impieghi, i quali risultano stranamente più stringenti sui prestiti concessi rispetto agli investimenti in derivati speculativi di secondo e terzo livello. Tale decisione non considera che tali strumenti finanziari sono di difficile valutazione in termini sia di corretta determinazione al *fair value* del loro valore iscrivibile in bilancio sia di incidenza del rischio sotteso alla effettiva e concreta recuperabilità

focalizzare le attenzioni sui crediti deteriorati introducendo stringenti regole contabili invece di porre limiti e vincoli agli investimenti su derivati, dove, peraltro, è più facile occultare perdite latenti, alterare le informazioni di bilancio e frodare i terzi risparmiatori. L'invocata diversa attenzione scaturisce anche dal differente peso valoriale in termini di rischio sistemico che i crediti deteriorati hanno nell'economia del sistema bancario europeo, dove questi ultimi ammontano, secondo i dati del trimestre 2018, a circa 820 miliardi di euro contro i 600.000 miliardi di euro di investimenti in derivati. Un'altra anomalia del sistema di regole europee è la centralità del patrimonio rispetto alla capacità reddituale, nel senso che si tende a valutare l'incidenza del capitale proprio sugli impieghi, omettendo di considerare la capacità dell'impresa

perché le imprese e le famiglie non riescono a pagare i loro debiti verso il sistema bancario. Un esame approfondito su questo tema farebbe comprendere la vera causa della crisi degli istituti di credito. Di fronte a questo problema sociale ed economico non mi sembra che l'Europa e i precedenti Governi abbiano introdotto misure idonee. Per non affrontare il vero problema della crisi bancaria sono stati, infatti, concessi finanziamenti a un tasso dello zero virgola alle banche e imposti livelli assolutamente alti di patrimonio rispetto agli impieghi; è stata introdotta inoltre la svalutazione crescente dei crediti deteriorati in percentuali definite e in in tempi contingentati entro i tre anni per i crediti *non performing loan* (NPL) privi di garanzia ed entro sette anni per quelli con garanzia reale. Queste ultime prescrizioni, del tutto sganciate dal contesto economico in cui l'impresa opera e dalla diversa efficienza territoriale del sistema di giustizia italiano, sono anch'esse ingiustificabili. Infine, la nuova riforma promossa dall'Unione europea sugli NPL sta determinando un altro importante fenomeno che potrebbe compromettere persino la sopravvivenza stessa del sistema bancario italiano. Trattasi della cessione di interi portafogli crediti in sofferenza a società finanziarie specializzate, prevalentemente internazionali. In conclusione, al di là delle cause che hanno inciso sulla situazione economico-finanziaria e sulla perdita dell'80 per cento di valore di Banca Carige, rimane discutibile l'intervento di commissariamento da parte di BCE sia per la perentorietà di applicazione di un regolamento europeo sia per i possibili effetti economici e giuridici anche di natura costituzionale che non mancherà di produrre. Sta di fatto che il sistema delle regole europee e dei controlli non ha permesso di evitare la crisi di una delle banche storiche italiane, la Carige, nata nel 1483. In venti anni, chi ci ha preceduto è stato capace di distruggere ciò che è stato costruito in sette secoli. Concludo questo mio breve intervento citando un passo del canto VI del Purgatorio del divino poeta, che, a proposito dell'occupazione dei popoli nordici sull'Italia, ebbe a dire: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello».

perché è importante avere un sistema creditizio in equilibrio, che non generi crisi. È utile a Genova e alla Liguria, perché Banca Carige è un primario attore di quel territorio. Si tratta di un decreto-legge che salva i correntisti e i loro risparmi; di un decreto che salva le imprese alle quali Banca Carige presta denaro; di un decreto che salva i lavoratori, non solo di Carige, ma anche delle aziende clienti di Banca Carige. Il provvedimento contiene due opzioni diverse per il futuro della banca. La garanzia per le passività di nuova emissione, prevista dall'articolo 1 del decreto Carige, ma prevista anche dall'articolo 1 del decreto per la tutela del risparmio fatto dal Governo Gentiloni e la ricapitalizzazione prudenziale, prevista dall'articolo 12 del decreto Carige in discussione, ma prevista anche, in forma identica, dall'articolo 13 del decreto-legge per la tutela del risparmio fatto dal Governo Gentiloni Le due opzioni di intervento hanno una diversa temporalità. La garanzia dello Stato prestata per le nuove emissioni obbligazionarie ci dice che, giustamente, è prioritaria la ricerca di una soluzione di mercato per la gestione dei problemi di Carige. Si tratta di un importante e forte messaggio che viene dato al Paese. Nessuno pensi che lo Stato possa correre a "mettere le pezze" dove altri hanno commesso degli errori. Certo, l'importanza di vedere tutelato il sistema creditizio impone allo Stato di intervenire con misure di aiuto ma, in prima battuta, questo aiuto si traduce in un sostegno all'iniziativa privata. Non si tratta di sostituirsi al privato. Quindi, al momento non c'è nessuna nazionalizzazione in cantiere.

occupati di crisi bancarie), quella della ricapitalizzazione prudenziale, non è affatto in contrasto con la soluzione privilegiata di mercato. Si tratta, anche in questo caso, di un messaggio chiaro, inviato a quanti sono interessati ad acquisire Carige, perché non si può negoziare all'infinito e giocare al tira e molla per contrattare sul prezzo di vendita. Per l'eventuale ricapitalizzazione statale, sappiamo tutti bene che sarebbe necessaria l'autorizzazione dell'Unione europea, perché l'eventuale intervento non si deve configurare come aiuto dello Stato vietato dalle norme europee. Proprio questa mattina, la commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, durante la sua audizione in Senato, ha affermato che le leggi contro gli aiuti di Stato esistono per dare sostegno alle banche, consentendo di mantenere la stabilità finanziaria, ma che l'altro obiettivo è fare in modo che la concorrenza fra le banche sia equa e che i contribuenti non finiscano per pagare un conto troppo salato. Un principio difeso in più di cinquecento casi in Europa, ha detto la Commissaria Dovendo quindi tenere aperta la porta per un intervento che necessiterebbe del beneplacito europeo, ed essendo chiaro che si tratta di un'eventualità che potrebbe, però, rendersi necessaria per dare corso alle positive ragioni a a sostegno del decreto-legge che richiamavo in apertura di questo intervento, dovendo quindi tenere aperta questa porta, mi permetto, signor Presidente, di dare un suggerimento alla maggioranza.

sono inutili gli insulti gratuiti presentati a istituzioni europee e a rappresentanti istituzionali europei; sono inutili i servizi giornalistici trasmessi dalla TV pubblica, che rendono indegna la televisione di Stato rispetto al ruolo che ha svolto a livello europeo e internazionale *(Applausi dal Gruppo PD)*. Dovremmo invece ricercare alleanze e non fratture con i *partner* europei, perché quando avremo bisogno di sostegno e di aiuto, nel momento in cui si dovesse verificare tale situazione, non dovremo trovarci nella condizione di ricevere sberle da chi è stato insultato da rappresentanti della maggioranza. il Partito Democratico ha fatto molto per tutelare il sistema creditizio, quindi i risparmiatori, i lavoratori e le imprese. La riforma delle banche popolari così come l'autoriforma del credito cooperativo hanno risposto all'esigenza strategica di consolidare la solidità patrimoniale del sistema creditizio proprio per poter meglio far fronte alle crisi sistemiche. Le crisi bancarie subentrate negli anni scorsi sono quindi state affrontate nell'ambito di questa strategia e anche la crisi di Carige è stata affrontata proprio con le medesime finalità e i medesimi presupposti. Carige si pone in totale continuità con le politiche sviluppate dai Governi del PD sulle crisi bancarie e sul sistema del credito. Abbiamo lo stesso identico quadro normativo, perché il decreto-legge Carige e quello sulle crisi bancarie sono esattamente identici; abbiamo la stessa direzione strategica, quella cioè di favorire le aggregazioni e le acquisizioni che rafforzino la solidità patrimoniale del sistema creditizio, la tenuta patrimoniale stessa e la capacità di smaltire le sofferenze. Abbiamo addirittura la stessa identica previsione di un possibile *bail in*, per quanto non auspicato ovviamente. Tuttavia l'articolo 20 del decreto-legge Carige, usando le stesse parole dell'articolo 22 del cosiddetto stabilisce che la ricapitalizzazione da parte dello Stato, cioè l'eventuale nazionalizzazione, potrà intervenire solo dopo l'applicazione di misure di ripartizione di ripartizione degli oneri, con l'obiettivo di contenere il ricorso a fondi pubblici. Come è noto, attraverso il *bail in* sono chiamati a pagare gli azionisti e gli obbligazionisti privilegiati delle banche e non la collettività con la fiscalità generale.

si degrada di uno scalino l'azione di risparmio che era stata acquistata dal risparmiatore in borsa, facendogli perdere i connessi vantaggi patrimoniali e aumentando invece di un gradino il rischio di azzeramento totale in caso di risoluzione della banca. Se ciò non bastasse, vengono convertite in azioni ordinarie anche le obbligazioni subordinate. Si tratta del cosiddetto *burden sharing*, una delle misure di *bail in* previste dalla normativa. Mi chiedo pertanto: dove sono le differenze

Avete presentato e votate un decreto-legge che, per strategie, quadro normativo e interventi, è esattamente identico a quanto avevamo prodotto noi e lo fate dopo che sui nostri provvedimenti avete scaricato vergognosi attacchi, dopo che ci avete vituperati violentemente, dopo che su alcuni dei nostri rappresentanti avete scaricato fango inutilmente! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Vi chiedo: con quale dignità voterete a favore di questo provvedimento, identico a quello che avevamo votato noi, quando sul nostro vi siete pronunciati in maniera vergognosa? Abbiate almeno la dignità di chiederci scusa per gli attacchi che ci avete rivolto e abbiate la dignità di chiedere scusa agli italiani per le falsità che avete loro raccontato.

dicendo che probabilmente questo argomento è talmente noto che non c'è necessità di parlarne.

è il fatto che, né il Governo del Partito Democratico - quando si è trovato a gestire le crisi di alcune banche - né l'attuale Governo hanno le hanno le idee chiare su come oggi devono essere gestite le crisi bancarie. Sono francamente un po' stufa di vedere cambiare il nemico a seconda della crisi bancaria di turno:

dobbiamo capire in che momento siamo, soprattutto sotto il profilo della valutazione della crisi economica, e individuare una strada.

il vice premier Di Maio era partito lancia in resta parlando di un decreto-legge che avrebbe salvato i risparmiatori, nazionalizzando la Carige.

Andatevi a vedere quello che hanno combinato con la truffa dei diamanti, per capire quello che riescono a fare ancora oggi le banche e gli intermediari. Non abbiamo però bisogno di *show*, da questo punto di vista.

chiara la scelta che si fa nel contesto di carattere economico e risparmiateci, possibilmente, le sceneggiate del "nemico": Commissioni d'inchiesta, azzeramenti, eccetera. Qui si tratta di salvare un territorio che si era agganciato a una banca di natura territoriale, tenendo conto del quadro generale dato dalla crisi di carattere economico.